L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

La seduta di oggi sarà sospesa fino alle ore 16 e riprenderà con l'informativa del Ministro dell'interno sui fatti occorsi in occasione di recenti manifestazioni di studenti relative alla morte del giovane Lorenzo Parelli. La discussione del decreto-legge sulla proroga dello stato di emergenza avrà inizio alle ore 9,30 di domani, con seduta senza orario di chiusura. La seduta sarà sospesa alle ore 13, in relazione agli adempimenti concernenti la cerimonia del Giorno del ricordo, che avrà luogo in Aula alle ore 16 con la presenza del Presidente della Repubblica. I lavori dell'Assemblea riprenderanno orientativamente alle ore 19. Resta confermata, se necessaria, la seduta di venerdì 11 fino alle ore 13. Il calendario della prossima settimana prevede l'eventuale seguito del decreto-legge sulla proroga dello stato di emergenza e, nella seduta di martedì 15 febbraio, la discussione di mozioni sul Nutri-score e il piano decennale From farm to fork. Mercoledì 16 saranno discussi i documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in materia di insindacabilità.

Signor Presidente, prima di avanzare la nostra proposta di calendario, vorrei brevemente spiegare perché si arriva a votare il calendario dei lavori non avendo ieri, in Conferenza dei Capigruppo, raggiunto la necessaria unanimità. L'unanimità non è stata raggiunta perché Fratelli d'Italia non condivide la proposta di un calendario peraltro astratto, perché ancora non sappiamo come si svolgeranno esattamente i lavori della Commissione di competenza - che vuole inserire uno scampoletto di tempo per giovedì sera. voglio essere chiara: non è naturalmente l'eventuale lavoro serale o notturno che ci spaventa. Quello che ci spaventa è il modo di procedere, che si potrebbe

a un'assenza di lavori della Commissione. Mi spiego: dovremmo discutere il disegno di legge n. 2488 di conversione del decreto-legge n. 221 cui l'emendamento del Governo ha aggiunto anche altri aspetti. Si tratta quindi di un atto importante che riguarda la materia sanitaria, la sorveglianza sanitaria e le tantissime misure di contenimento dell'epidemia. La Commissione La Commissione è stata convocata e sconvocata più di una volta e fondamentalmente non ha ancora cominciato i suoi lavori, al di là della discussione generale. A noi di Fratelli d'Italia non piace piace fare e disfare il calendario in base al criterio della fretta, piegando gli orari che servono alla discussione e al confronto per alcune esigenze che non mettono al primo posto, come invece dovrebbe essere fatto, l'importanza dei provvedimenti e anche la funzione di quest'Assemblea. La questione, in sintesi, non è certamente

di distanza dalle parole di richiamo del presidente Mattarella pronunciate durante il secondo giuramento, e mi riferisco in particolare all'espressione di non comprimere e non dilatare i tempi di discussione in Aula, che poi concettualmente è un principio sano e sacrosanto... *(Brusio).* Chiedo ai colleghi della Lega se possono fare silenzio, perché si tratta solo di un minuto. Grazie per l'attenzione così cortese. Dicevo che si tratta di difendere il principio della centralità del Parlamento. Il decreto-legge è molto importante, merita tempi e modi di discussione e lo meritano anche i numerosi emendamenti, può puntare sullo scampoletto di tempo di giovedì sera. Posso anche immaginare il modo frettoloso in

depositate al tavolo della Presidenza e non discusse in Assemblea *(Applausi)*, accompagnate addirittura da un applauso liberatorio, con la rinuncia quindi a svolgere una funzione. Sono discorsi che poi arrivano all'esterno, perché non siamo in una bolla e non ci vogliamo finire. Pensiamo quindi che questa ipotesi di rimaneggiamento del calendario vada a vantaggio delle esigenze di chi vuole tornare a casa e non della

Penso che chi non è interessato possa tranquillamente uscire e tornare per il voto. Come dicevo, purtroppo non è la prima volta che dobbiamo subire questa - se la vogliamo chiamare elegantemente - asistematicità. Penso, ad esempio, ai tempi di discussione e di approvazione

una nuova finestra"). L'ordine del giorno reca: «Informativa del Ministro dell'interno sui fatti occorsi in occasione di recenti manifestazioni

Signora Presidente, onorevoli senatori, prima di riferire sugli episodi oggetto dell'informativa odierna, desidero rinnovare, da parte di tutto il Governo e mia personale, il cordoglio

che con l'impegno e la freschezza dei suoi diciotto anni testimoniava la determinazione del nostro Paese a rialzarsi dalla crisi devastante indotta dalla pandemia. Sono proprio i giovani ad aver risentito più intensamente delle restrizioni sociali, delle diseguaglianze, delle marginalità e delle occasioni mancate che sono alla base di un malessere profondo, non sempre compreso. Più voci autorevoli si sono soffermate recentemente sulla profondità di questa crisi, dovuta anche al mancato ascolto da parte degli adulti in un quadro di angoscia esistenziale che ha cambiato i nostri comportamenti, creando distanze umane sconosciute e incidendo profondamente sulla nostra società. Così, la morte inaccettabile di un giovane, per giunta in un momento che avrebbe dovuto essere di massima sicurezza perché collocato nell'ambito di uno *stage* curricolare, ha originato manifestazioni di solidarietà e proteste da parte dei suoi coetanei. È innegabile che ognuno di noi abbia provato sentimenti di incredulità e sgomento, così come è indubitabile che queste proteste giovanili esprimano anche la voglia di partecipazione di un mondo che durante la pandemia ha sofferto in particolar modo l'isolamento. È comunque un segno di vitalità della nostra democrazia che ci fa ben sperare nel futuro. D'altro canto, però, la democrazia ha le sue regole, dalle quali non si può prescindere mai, soprattutto quando si tratta di regole poste a presidio del cruciale bilanciamento dei valori costituzionali, quali il diritto di manifestare liberamente e la tutela della salute pubblica. E qui vengo ai fatti. A seguito della morte di Lorenzo, avvenuta il 21 gennaio scorso a Lauzacco, in provincia di Udine, hanno avuto luogo diverse manifestazioni studentesche volte a commemorare il giovane e a contestare le modalità di svolgimento delle attività di formazione al lavoro inserite nel percorso didattico. A tali finalità si è poi aggiunta la protesta nei confronti del ripristino dello svolgimento delle prove scritte in occasione dei prossimi esami di maturità. Una prima manifestazione estemporanea e non ritualmente preavvisata si è svolta a Roma il 23 gennaio per iniziativa del movimento studentesco La Lupa, facendo registrare la partecipazione di altri sodalizi come la Opposizione studentesca d'alternativa (OSA) e il Fronte della gioventù comunista, per una presenza complessiva di circa 200 persone. sede far presente che le attività informative di polizia avevano fatto emergere la precisa intenzione di alcuni partecipanti, appartenenti ai centri sociali capitolini e aderenti a gruppi di matrice anarchica, di trasformare la stessa manifestazione in un'occasione di scontro fisico con la polizia. In effetti, nonostante sia stato svolto in quella circostanza più di un tentativo di mediazione e siano stati rivolti ripetuti inviti a desistere, un gruppo di manifestanti, staccandosi da piazza della Rotonda, luogo d'incontro dei partecipanti, si è mosso in corteo, contravvenendo così alle vigenti disposizioni introdotte per finalità anti-Covid, fino ad impattare con lo schieramento di polizia disposto a protezione di obiettivi sensibili. L'intenzione di arrivare ad uno scontro con i rappresentanti delle Forze dell'ordine era testimoniata anche dal travisamento di alcuni dei manifestanti con caschi, cappucci e soprattutto dal ripetuto lancio di fumogeni e bombe carta contro gli appartenenti alle Forze dell'ordine, alcuni dei quali raggiunti da calci e pugni, tanto che alla fine della giornata, tra gli operatori di polizia contusi, quattro hanno dovuto far ricorso a cure mediche. Non si hanno notizie ufficiali sul numero dei contusi tra i manifestanti, ma risulta che uno di loro ha sporto denuncia per lesioni all'autorità giudiziaria. Per concludere la mia esposizione sui fatti di Roma, informo che tre dimostranti sono stati denunciati, ai sensi dell'articolo 18 del testo unico di pubblica sicurezza (TUPS), per il mancato preavviso della manifestazione e che sono tutt'ora in corso indagini con l'ausilio della Polizia scientifica. Il 28 gennaio il Fronte della gioventù comunista ha indetto sugli stessi temi una manifestazione studentesca a carattere nazionale, articolata su 35 manifestazioni, 31 delle quali si sono svolte regolarmente. A Milano, Torino, Roma e Napoli si sono invece verificati episodi critici sotto il profilo dell'ordine pubblico, dei quali ora dirò. La manifestazione milanese, indotta dal coordinamento collettivo e studentesco, era stata preannunciata in forma di presidio statico presso piazza Missori e via Pantano. Secondo gli organizzatori, avrebbe dovuto vedere la partecipazione di circa 100 persone, ma in realtà si è poi arrivati a circa 300. Un'ora dopo l'inizio della manifestazione, ossia intorno alle ore 16,30, i dimostranti, violando anche in questo caso le disposizioni anti-Covid, abbandonavano la piazza per dirigersi compattamente in corteo verso la vicina sede di Assolombarda, a protezione della quale era stato disposto uno schieramento dei reparti mobili. Un consistente gruppo di manifestanti, circa 50, rimuoveva le transenne ivi collocate e, nel tentativo di aprirsi a forza un varco verso la sede di Assolombarda, entrava in contatto con gli operatori di polizia, seguivano il lancio contro questi ultimi di uova contenenti vernice rossa e l'accensione di fumogeni. Il protrarsi di tale accesa fase di confronto ha comportato l'effettuazione di due brevi azioni di alleggerimento,

Gli elementi più facinorosi sono stati individuati dalla questura in alcuni esponenti del Coordinamento collettivi studenteschi, attualmente legato al «Centro sociale Cantiere» nonché in soggetti appartenenti all'area antagonista e anarchica. Sulla base di questa prima attività di indagine, cinque attivisti dei movimenti studenteschi sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, mentre uno di questi è stato anche deferito per la violazione dell'articolo 18 del testo Al termine della manifestazione due operatori del reparto mobile di Milano hanno riportato lievi escoriazioni, mentre tra i manifestanti si sono contati taluni contusi, di cui uno è rimasto ferito al capo e ha peraltro rifiutato l'intervento del personale sanitario. Da successivi accertamenti svolti presso i locali nosocomi, non risultano manifestanti refertati. Passo ora alla manifestazione di Torino che, come quella di Milano, era stata preannunciata per la mattina del 28 gennaio in forma statica; soggetto promotore il collettivo studentesco Fronte della gioventù comunista; luogo di convegno piazza Arbarello, dove si sono radunate circa 300 persone, tra cui, insieme ad appartenenti a vari collettivi studenteschi e ad esponenti degli ambienti antagonisti e anarchici torinesi, erano presenti numerosi militanti del noto centro sociale Askatasuna, espressione locale del movimento di Autonomia operaia, particolarmente attivo su diversi temi e distintosi in particolare per azioni ed episodi criminosi commessi nel corso di manifestazioni, occupazioni, sgombri di stabili, occupati abusivamente, ovvero per altri episodi di rilievo penale. Preciso che gli organizzatori avevano inizialmente chiesto di effettuare un corteo e che dopo un chiarimento con la questura, circa i vincoli imposti dalla normativa sul Covid in zona arancione, la manifestazione era stata trasformata in un presidio fisso. Ciononostante un consistente gruppo di partecipanti muoveva in corteo contro lo schieramento delle Forze dell'ordine posto a chiusura della piazza, cercando più volte di rompere lo sbarramento. L'azione si è svolta in pochi minuti e ha riguardato i vari punti di dispiegamento del dispositivo di polizia presente nella piazza. In tali frangenti, si sono verificati momenti di elevata tensione, dovuta al contatto fisico tra i dimostranti più accesi e il personale del reparto mobile. Dopo aver inizialmente utilizzato gli scudi in dotazione, gli operatori della polizia, a causa dei violenti tentativi di sfondamento esercitati con calci e pugni, hanno fatto ricorso ad azioni di respingimento e a un intervento di alleggerimento, in quest'ultimo caso anche con l'impiego dello sfollagente, ottenendo l'arretramento del fronte dei dimostranti. L'azione non ha avuto, tuttavia, l'esito di disperdere i manifestanti, che continuavano pertanto a premere sullo schieramento di pubblica sicurezza per altre due ore, durante le quali si susseguivano repentini spostamenti di gruppi organizzati di manifestanti, accompagnati dal lancio di pietre e di bottiglie di vetro, cui hanno corrisposto ulteriori interventi delle Forze di polizia. Il bilancio dei feriti è il seguente: un operatore del reparto mobile, colpito al volto da un pugno, ha riportato una prognosi di cinque giorni; otto sono, invece, i manifestanti medicati sul posto, mentre altre 10 persone hanno fatto ricorso a cure mediche presso i principali ospedali cittadini, riportando prognosi fino a un massimo di dodici giorni. I primi risultati investigativi, frutto delle attività condotte dalla DIGOS con l'ausilio di tutte le immagini disponibili, comprese quelle reperite sul *web*, attestano che gli scontri avvenuti nella manifestazione di Torino hanno visto all'opera, con un preciso ruolo di regia, militanti di Askatasuna. delle 17 persone denunciate all'autorità giudiziaria per vari reati, tra cui resistenza aggravata a pubblico ufficiale, sono noti attivisti del predetto centro sociale, mentre gli altri quattro sono rappresentanti dei vari collettivi studenteschi. Venendo ora alla manifestazione di Roma, preciso che l'iniziativa è stata assunta dallo stesso movimento studentesco La Lupa, che aveva indetto la precedente manifestazione del 23 gennaio. Durante l'evento, cui hanno partecipato circa 500 persone, un gruppo di manifestanti si è reso responsabile di un fitto lancio di pietre e bottiglie, fumogeni e altri oggetti contundenti contro le Forze di polizia. Non essendosi verificato, tuttavia, alcun tentativo di sfondamento ed essendo quindi mancato ogni contatto fisico tra le Forze dell'ordine e i facinorosi, non vi è stata la necessità di ricorrere a interventi coattivi. La manifestazione si è conclusa registrando un ferito tra gli operatori di polizia, il quale ha riportato lievi escoriazioni per l'esplosione di una bomba carta. Riferisco, infine, sui fatti avvenuti a Napoli. Anche in questo caso, la manifestazione ha visto l'aggressione di soggetti estranei al movimento studentesco, essendosi evidenziata la presenza di appartenenti a centri sociali e al sodalizio "Disoccupati 7 novembre". Il luogo di concentrazione dei partecipanti, circa 250, era stato individuato nella centralissima piazza dei Martiri, dove è ubicata la sede dell'Unione degli Industriali, per accedere alla quale i dimostranti hanno tentato di forzare il dispositivo di polizia, dopo aver dato fuoco ad alcuni fumogeni e lanciato in direzione della predetta sede palloncini di vernice colorata. È stata necessario pertanto un'azione di alleggerimento, allo scopo di disperdere i manifestanti, i quali poi hanno dato luogo a un corteo, svoltosi senza alcun incidente. Non ci sono stati feriti, né tra dimostranti né tra le Forze di polizia. Il tentativo di rompere lo sbarramento di sicurezza ha portato al deferimento all'autorità giudiziaria di quattro manifestanti, tre dei quali appartenenti ai centri sociali e al citato movimento "Disoccupati 7 novembre". Questo è solo il risultato delle prime attività investigative, essendo ancora in corso ulteriori accertamenti volti a individuare altri possibili autori delle condotte violente. Nell'esprimere la mia solidarietà agli operatori di polizia rimasti contusi in occasione degli scontri, sui quali ho appena riferito, preciso che l'intera documentazione visiva, sia quella ripresa dalla Polizia scientifica, sia quella acquisibile da fonti aperte, è stata messa immediatamente a disposizione dell'autorità giudiziaria, come accade in tutti i casi in cui, nel corso di manifestazioni pubbliche, avvengano fatti integranti ipotesi di reato. La magistratura inquirente, pertanto, è nelle piene condizioni di accertare la dinamica dei fatti e le responsabilità connesse a tali accadimenti, comprese quelle eventualmente riconducibili alla condotta degli operatori di polizia. Signora Presidente, onorevoli senatori, alla ricostruzione dei fatti accaduti il 28 gennaio scorso vorrei aggiungere alcune considerazioni conclusive: come già affermato in altre circostanze in cui ho avuto modo e occasione di riferire in Parlamento, la difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica in un ordinamento democratico richiede puntuale esercizio delle responsabilità di ciascuno; prudente apprezzamento delle circostanze e senso della misura, saldamente inquadrati nella cornice di criteri unitari e non discriminatori, premessa indispensabile per garantire in ogni situazione il bilanciamento dei diversi valori costituzionali in gioco. È in quest'ottica che sono state affrontate - per fare un esempio - le circa 5.000 manifestazioni svoltesi l'anno scorso contro il *green pass* e le misure restrittive anti-Covid; solo 115 delle quali hanno fatto registrare turbative, con un impegno davvero rilevante delle Forze di polizia, chiamate a far rispettare ogni giorno regole fondamentali per il corretto e sereno svolgimento della vita civile e democratica della nostra comunità nazionale. Ed è anche in omaggio a questo impegno che chi ai diversi livelli è chiamato a esercitare responsabilità istituzionali e operative, connesse alla salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, deve riflettere a fondo quando in questo difficile lavoro si verificano fatti incresciosi, come quelli che il 28 gennaio scorso hanno causato conseguenze a danno di alcuni giovani studenti estranei ai gruppi dei facinorosi presenti nelle piazze e, tuttavia, rimasti coinvolti nei tafferugli. Come ho accennato all'inizio, non possiamo non vedere come la protesta degli studenti nasca anche da un forte disagio originato dalle restrizioni della pandemia, che hanno finito per comprimere il mondo dei giovani nella loro dimensione formativa e aggregativa. Abbiamo tutti il dovere di comprendere e di disporci all'ascolto di fronte a una realtà, quella giovanile, divenuta ancora più complessa a causa degli inediti problemi che l'emergenza sanitaria ha portato con sé. Ce lo ha ricordato qualche giorno fa anche il Presidente della Repubblica, affermando che è doveroso ascoltare la voce degli studenti che avvertono tutte le difficoltà del loro domani e cercano di esprimere esigenze e domande volte a superare squilibri e contraddizioni. La via maestra è il confronto. Lo sforzo che occorre fare, soprattutto quando le cose non vanno per il meglio, è cercare di individuare modalità più idonee per contemperare il diritto a manifestare con il dovere delle Forze di polizia di far rispettare la legge. Le stesse norme vigenti, del resto, prevedono che gli organizzatori e gli uffici delle questure possano dialogare, affinché l'evento si svolga senza malintesi, dai quali possono scaturire tensioni difficilmente gestibili sul piano dell'ordine pubblico. L'ho ricordato anche in una mia recente direttiva in materia di manifestazioni pubbliche, adottata a novembre del 2021, con la quale ho espressamente richiamato l'applicazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza nella modulazione delle misure interdittive e prescrittive. Il 4 febbraio scorso, nelle stesse grandi città interessate dai fatti del 28 gennaio (Milano, Torino, Roma, Napoli, così come in altre significative realtà italiane), le manifestazioni studentesche si sono svolte senza generare criticità raffrontabili con quelle su cui oggi ho riferito. Al conseguimento di questo risultato si è giunti grazie a una moderazione del livello di protesta e in virtù di un intenso dialogo tra la componente studentesca e le autorità preposte alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Nella mia esperienza professionale ho avuto modo di verificare sul campo come flessibilità ed equilibrio siano caratteristiche e qualità di tutte le Forze dell'ordine italiane e sono certa che sapranno farne il più ampio uso ogni volta che la situazione lo richiederà. Ne sono certa e per questo ho fiducia in loro. Allo stesso tempo ho ben chiaro che il livello complessivo di efficacia del loro operato dipende in misura non secondaria dalla qualità delle dotazioni tecniche a loro disposizione, da quelle che hanno come fine la tutela dell'incolumità degli operatori fino ai dispositivi che garantiscono la trasparenza della loro attività e rendono sempre possibile ricostruire l'esatto andamento dei fatti. Mi riferisco qui alle telecamere di cui sono state recentemente dotate le Forze di polizia (la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri), denominate *bodycam*, che verranno usate dagli operatori impegnati nei servizi di ordine pubblico. L'utilizzo di tali nuove apparecchiature avverrà nel pieno rispetto delle direttive impartite dal Garante della *privacy*, che ha definito le procedure di attivazione nonché le regole sull'uso delle registrazioni e la conservazione delle immagini. Credo si tratti di un passo importante, destinato a rinsaldare ulteriormente i sentimenti di vicinanza e affetto che legano i cittadini italiani alle Forze di polizia, garanti della difesa delle libertà civili sancite dalla Costituzione della Repubblica.

la responsabilità del sangue e delle teste degli studenti minorenni spaccate dai manganelli della Polizia di Stato ricade integralmente su di lei, senza possibilità di scusa alcuna. Lei dice che tra i manifestanti e tra gli studenti si nascondevano agitatori. Nessun agitatore, se non gli agenti provocatori che sempre più spesso vediamo nelle piazze, noi abbiamo potuto ravvisare; quegli agenti provocatori che sono funzionali, prima, alla repressione dura e sanguigna in piazza e che le consentono, dopo, di adottare i provvedimenti per limitare il dissenso e impedire i cortei. Peraltro, sono gli stessi agenti provocatori che, una volta colti dalle telecamere, lei giustifica con le famose frasi sulle «forze ondulatorie», con cui si è coperta anche di ridicolo. Ministro Lamorgese, il suo operato e l'operato del Governo di cui fa parte si stanno connotando sempre di più per obiettivi, modalità esecutive e propaganda che sono proprie dei regimi autoritari. Pertanto, in questo luogo di rappresentanti del popolo, ho il dovere di farle sentire il peso dello sdegno e del disprezzo che un popolo, che non avrà

Signor Presidente, in primo luogo voglio ringraziare la ministra Lamorgese per essere venuta qui a rendere l'informativa sui gravi fatti degli scorsi giorni. Credo sia indispensabile chiarire i profili di criticità che certamente sono emersi dalla gestione della manifestazione di studenti dei giorni scorsi, indetta per la tragica morte del giovane Lorenzo Parelli. Mi preme fin da subito operare una premessa. Nonostante questi accadimenti, non si può mettere in discussione il ruolo fondamentale che le Forze di polizia rivestono nell'assicurare quotidianamente il pieno svolgimento della democrazia; il loro operato è essenziale e rassicurante per l'intera collettività. La loro dedizione e il loro senso delle istituzioni si sono manifestati in tutta la loro pregnanza anche e soprattutto durante i lunghi anni di emergenza sanitaria. è proprio sulla scorta di questi sentimenti sinceri di gratitudine che noi tutti nutriamo nei confronti delle Forze dell'ordine che stupiscono ancora di più i fatti dei giorni scorsi. Siamo rimasti sgomenti di fronte ai volti dei ragazzi che hanno partecipato alla manifestazione; ragazzi malmenati e spaventati. allora difficile capire perché si è avvertita la necessità di reprimere in maniera così violenta manifestazioni spontanee di studenti che, dopo anni difficili di torpore e di asocialità forzata dovuta alla pandemia, sono scesi in piazza per esprimere solidarietà nei confronti di un giovane che ha tragicamente perso la vita durante l'orario l'orario scolastico. Mi hanno molto colpito le parole della mamma del giovane Lorenzo, che ha definito come una carezza le manifestazioni dei giovani per suo figlio. Credo che quella carezza non possa e non debba assumere i tratti della violenza. Le misure volte a tutelare l'ordine pubblico, anche se si tratta di misure più stringenti dettate dalle esigenze di contenere la pandemia e dalla salvaguardia della sicurezza pubblica, devono essere sempre bilanciate con la tutela del diritto costituzionalmente garantito alla manifestazione di pensiero. La risposta a tutela dell'ordine pubblico non può che essere sempre proporzionata e guidata da un bilanciamento. Lei, signora Ministra, in questi giorni ha parlato di un cortocircuito del sistema, che è esploso con violenza quando le Forze di polizia si sono trovate di fronte a persone che volevano manifestare in zone non previste. Ovviamente, le singole responsabilità di chi ha fatto un uso sproporzionato e non necessario della violenza saranno accertate. Tuttavia, in questa sede occorre respingere con forza un simile *modus operandi*. Non possiamo e non dobbiamo permettere che simili episodi possano accadere nuovamente. E non possiamo farlo non solo perché ciò si traduce in una risposta totalmente sproporzionata di fronte alla manifestazione di pensiero, ma anche per la stessa credibilità e serietà delle Forze dell'ordine. Ciò emerge ancora di più nelle manifestazioni studentesche, dove ci sono giovani che desiderano semplicemente far sentire la propria voce. Credo che in questo caso ci sia una valenza ulteriore: i giovani sono stati proprio la categoria generazionale più colpita dalla pandemia. Due anni scolastici in DAD e una socialità fortemente ridotta hanno più che mai mostrato le fragilità e le debolezze dei più giovani, che hanno dovuto costruire un nuovo modo di fare scuola e una nuova modalità di interfacciarsi con gli altri. L'impatto delle violenze dei giorni scorsi diventa allora più assordante se lo caliamo nel contesto attuale. Gli studenti che sono scesi in piazza chiedono una corretta applicazione dell'istituto della alternanza scuola-lavoro e la previsione di regole certe che segnino la fondatezza di quel tempo di quel tempo impiegato altrove rispetto ai banchi di scuola. Ebbene, come rappresentanti delle istituzioni abbiamo il dovere di ascoltare, e non solo per evitare altri episodi di repressione violenta, ma anche e soprattutto perché il nostro compito è dedicarci a quanto accade nel mondo giovanile e raccogliere le loro istanze. La scuola ha un compito alto, che è la formazione certamente di persone preparate da un punto di vista culturale; persone mature e consapevoli delle proprie capacità e in grado di esprimerle; persone responsabili. non credo che questo modo di intendere la scuola sia incompatibile con il mondo del lavoro; anzi, credo che lo completi. La scuola può avere un ruolo fondamentale nel trasmettere conoscenze più propriamente tecniche e pratiche. Lo può fare fungendo da ponte per il mondo del lavoro, fornendo ai ragazzi la possibilità di saggiare con mano ciò che li aspetta dopo qualche anno. L'alternanza scuola-lavoro è un istituto che nasce dieci anni fa, ma che può ancora funzionare bene se si valorizzano i percorsi formativi.

Dobbiamo fare tutto in piena sicurezza. Signor Presidente, concludo. Pensiamo a migliorare questo istituto, pensiamo a riformarlo e poniamoci in atteggiamento di ascolto nei confronti dei più giovani. La morte di Lorenzo sia sempre ricordata come monito perché ogni lavoro, di qualsiasi tipo, a tempo determinato o indeterminato, sia sempre svolto nel massimo rispetto dei sistemi di sicurezza. *(Applausi)*.

invece è venuta qui a parlare di un concetto: l'impunità, la vostra impunita. Qui non si tratta di un singolo caso. Lei è diventata un rappresentante di uno Stato che ha un atteggiamento paradigmatico, che noi cerchiamo di sovvertire inutilmente. Lei è rappresentante di uno Stato che si fa forte con i deboli e debole con i forti: forti: è la realtà di questa modalità. *(Applausi).* La mamma di Lorenzo Parelli ha detto che gli studenti in piazza sono stati una carezza per suo figlio, che non stava riprendendosi da un periodo difficile, entusiasta di lavorare; stava semplicemente facendo l'alternanza scuola-lavoro perché era obbligato a farla, e non perché entusiasta di farlo, come ha detto lei. E invece lo Stato cosa ha fatto agli studenti a cui la mamma del ragazzo voleva mandare una carezza? Li ha picchiati selvaggiamente, senza pietà, e le telecamere hanno mostrato una violenza inaudita verso dei minorenni che sono finiti in ospedale, Ministro, e lei è responsabile di questo. altre alte cariche dello Stato. Non possiamo sempre scaricare sulla Polizia di Stato le responsabilità di una gestione inadeguata della sicurezza, perché questa è la realtà. Lei ha parlato di infiltrati; ha parlato di chissà quali potenziali pericoli che invece sono stati smentiti dalle telecamere; ha parlato anche di un corto circuito con i ragazzi, perché non possiamo ignorare che in questo momento c'è una circolare per la salute pubblica. A novembre, però, da un palco di una manifestazione no *green pass* è stato annunciato l'assalto alla CGIL, e anche lì c'erano delle restrizioni di salute pubblica, e invece siete rimasti a braccia conserte accompagnato manifestanti violenti a demolire la sede di un sindacato *(Applausi)*, nella totale indolenza delle dirigenze e delle Forze dell'ordine presenti. Ministro, lei ha detto anche che i codici identificativi delle Forze dell'ordine non servono perché ci saranno le telecamere sulle divise. La informo che una cosa non esclude l'altra: possiamo avere sia i codici che le telecamere. In secondo luogo, certamente le telecamere sono una garanzia in più, ma con i codici si dà la possibilità ai cittadini di denunciare senza impedimenti burocratici. Soprattutto, a lei che vuole tutelare le Forze dell'ordine, faccio presente che questi atteggiamenti vanno a detrimento di quegli agenti di polizia che indossano la divisa con onore, fanno bene il proprio lavoro e finiscono in pronto soccorso per la gestione indegna da parte degli agenti provocatori. Quindi, lei è responsabile sia dei ragazzi feriti sia dello stigma che si portano addosso quegli agenti che lavorano bene. La informo che Amnesty International ha portato al Viminale 155.000 firme per introdurre i codici identificativi delle Forze dell'ordine ed esistono proposte di legge, depositate alla Camera come al Senato già nella scorsa legislatura, in attesa di essere discusse. Il gioco al rilancio che fa lei con le telecamere, parlando parlando male di queste proposte di legge, serve solo a perdere tempo. Approviamo subito la norma per i codici identificativi prodotta anche da Amnesty International, che magari di diritti umani ne sa un pochino di più di questo Stato e di questo Governo che invece li offende e li umilia. quindi due ordini di problemi. Il primo è che una divisa indossata con onore e responsabilità non può essere utilizzata da alcuni come scudo per le proprie responsabilità e i propri gesti; a questo si pone un rimedio con i codici identificativi. Il secondo è il concetto di impunità: non ho riscontrato, da parte sua,

Ribadiamo in questa sede il nostro cordoglio alla famiglia, agli amici di Lorenzo, ai compagni di scuola dell'Istituto salesiano «Bearzi» di Udine e a tutta la comunità di cui lo studente faceva parte. Oggi, però, credo che sia nostro dovere approfondire aspetti che la tragica morte di Lorenzo ci suggerisce: uno di questi è il tema della utilità della ex alternanza scuola-lavoro - ora si chiama in maniera diversa - o, come nel caso di o, come nel caso di Lorenzo, dei percorsi di apprendimento duale o di tutta la galassia dei tirocini. È nostro dovere chiederci se la riforma Moratti che l'ha istituita nel 2003, e che poi è stata resa strutturale dal Governo Renzi, abbia centrato il suo obiettivo, che era quello di creare un ponte tra l'apprendimento didattico e quello pratico per favorire l'orientamento dei ragazzi, per offrire agli studenti e alle studentesse competenze utilizzabili fin da subito sul mercato del lavoro; il tutto basato sul presupposto che si possa imparare e acquisire conoscenze sia a scuola, sia in azienda. I risultati di questi anni non sono particolarmente soddisfacenti per diversi motivi: ad esempio, non tutti i luoghi di lavoro e le aziende possono avere una valenza formativa significativa; i *tutor* aziendali a volte non sono all'altezza della situazione e del difficile compito; non tutte le aziende sono capaci di trasmettere competenze e formazione, specialmente quelle aziende che già di formazione ne fanno poca o nulla per i propri dipendenti. Devo anche rimarcare quei casi in cui si utilizza questo istituto per sostituire manodopera salariata con studenti a costo zero o quasi zero. Noi crediamo che la scuola e l'istruzione in generale abbiano un compito ben più alto della mera preparazione al lavoro, ma debbano essere motore di inclusione sociale, di consapevolezza culturale, di sviluppo di coscienze di individui, di promozione di rapporti virtuosi tra l'individuo e la comunità, perché è grazie alla scuola che possiamo comprendere i diritti, ma anche i doveri di ciascun cittadino e il suo ruolo nella società.

non di sfruttamento di giovani studenti. Il Paese ha diverse necessità e noi mettiamo al centro dei nostri sforzi il miglioramento della scuola, dell'istruzione, della ricerca come uniche possibilità di sviluppo sociale ed economico. *(Applausi)*. queste fasi di formazione e di preparazione al lavoro devono avvenire in piena sicurezza e purtroppo il caso di Lorenzo evidenzia una situazione che sicuramente non è ottimale per quanto riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro, che è poco attenzionata nel nostro Paese, atteso che oggi registriamo una media di quasi quattro morti al giorno nelle aziende, nelle fabbriche, nei cantieri. L'altro aspetto su cui dobbiamo riflettere è connesso alle manifestazioni dei giovani che protestavano per la morte assurda di Lorenzo e per affermare che è assolutamente inaccettabile che uno studente sia messo in pericolo di vita mentre fa formazione. Questo ci dice che i nostri giovani nati nel nuovo millennio costituiscono una generazione cosciente del proprio ruolo e che vuole partecipare al dibattito pubblico, pretendendo giustamente i propri spazi. A questo proposito, devo rimarcare che le scene di forte

nostri giovani - ragazze e ragazzi - con la testa spaccata dalle manganellate. Noi confidiamo nel suo lavoro, ma riteniamo davvero necessari...

Sappiamo bene che questa è una generazione che potremmo definire dei tanti Telemaco, a cui per due anni è stato impedito anche solo di guardare l'orizzonte,

non rabbia. Questi ragazzi - come è stato ben ricordato prima - sono scossi dalla perdita di un ragazzo come loro, Lorenzo Parelli la morte più bianca e innocente, se è possibile quantificare l'intollerabilità di perdere la vita in quel modo hanno bisogno di ritrovare la voce per manifestare il vuoto di fiducia e futuro che sentono, con un disagio accresciuto dai durissimi anni passati. essi andavano un po' più accompagnati e controllati per la sicurezza loro e di tutti i cittadini. Abbiamo però compreso, signora Ministra - come lei ha ben spiegato - l'esigenza di contenimento che è propria di chi gestisce l'ordine pubblico, e di questo ringraziamo le Forze dell'ordine che compiono il loro dovere, senza risparmiarsi, a tutela di tutti noi. Contemporaneamente, però, questi ragazzi vanno ascoltati perché nelle manifestazioni è accaduto comunque un evento positivo: una rinnovata presa di coscienza, una ritrovata vitalità, una ritrovata voglia di partecipazione della generazione che più di tutte ha pagato il prezzo del Covid. Si tratta di un prezzo altissimo che i più giovani hanno pagato con la chiusura della scuola della scuola che noi di Italia Viva, per primi, abbiamo chiesto di riaprire durante la prima ondata. La scuola è il primo presidio di normalità e per tutto il tempo abbiamo lavorato e ottenuto di tenerla viva e in presenza. La scuola è il cuore della società e senza di essa non c'è niente e il mondo si ferma. ferma. È arrivato - lo stiamo dicendo tutti - il momento di tornare alla normalità. Il Governo sta predisponendo le misure che gradualmente ci permetteranno di ridurre le restrizioni. Però normalità significa anche recuperare la ritualità della partecipazione sociale e politica alla costruzione di una coscienza comune; e certo non possiamo fare a meno proprio di queste voci, delle voci dei più giovani.

nel cui nome e ricordo gli studenti erano scesi in piazza, certamente con una piattaforma variegata, non sempre condivisibile, come nel caso dello scritto alla maturità, ma comunque espressione di quella ritrovata normalità che tanto desideriamo e per la quale ci adoperiamo. È finita, purtroppo, con alcuni volti tumefatti di ragazzi minorenni che forse non avremmo voluto vedere e che sicuramente hanno fatto male. Ma sono certa che, se ci sono state delle responsabilità personali, queste saranno accertate. Lei ha parlato di possibili infiltrati in piazza

è giusto fare chiarezza subito e farla fino in fondo. Lo dobbiamo anche ricordando chi non c'è più, come Lorenzo. Grazie, signora Presidente; grazie, signora Ministra.

Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, innanzitutto lasciatemi dire che naturalmente Fratelli d'Italia si stringe intorno alla famiglia di Lorenzo, perché tutti siamo genitori e ne capiamo il dolore, il dramma. Perdere un figlio nell'orario di scuola, perdere un figlio nel programma scolastico scuola-lavoro impone a ognuno di noi

Ministro Lamorgese, è evidente che lei ha difficoltà a gestire l'ordine pubblico. Ho ascoltato con attenzione la sua informativa, scritta dai suoi uffici, dove c'è prima la descrizione delle manifestazioni. Ma si è dimenticata di dire la cosa più importante: lei, signor Ministro, non è stata in grado di dividere gli studenti, coloro che erano in piazza a manifestare per una causa giusta, come la morte del loro amico, del loro studente, dai centri sociali, dai provocatori, dagli infiltrati. Vede, signor Ministro, il suo compito dovrebbe essere quello di prevenire e di che in queste piazze a pagare non siano gli studenti, perché quelle facce piene di sangue ricadono sul suo operato, signor Ministro. Il fatto di mettere le Forze dell'ordine, in balia di tutti e di nessuno è una sua responsabilità, perché lei è al vertice di quel Ministero, è l'anello ultimo della catena di comando. comando. È inutile che oggi, oltre alla sua incapacità e al suo immobilismo, ci venga a far percepire che in fondo poi un capro espiatorio lo troverà. Ma non lo dovrà trovare nelle Forze dell'ordine, che noi difendiamo e difenderemo sempre per il loro operato. Le Forze dell'ordine fanno capo a lei, signor Ministro, ed è lei che ne ha la responsabilità. Anche questa volta le manifestazioni le sono scappate di mano, perché non ha saputo prevenire. Che ci siano i centri sociali, che ci siano i provocatori in ogni manifestazione è ormai evidente; l'abbiamo visto nelle manifestazioni contro il *green pass*, dove c'erano le famiglie con i passeggini, ma c'erano anche i centri sociali e gli infiltrati. *(Applausi)*. E la sua risposta qual è? Lei fa sempre e comunque di tutta l'erba un fascio; questo non è più possibile. più possibile. Signor Ministro, se fossimo in altri Stati, in Francia, nel Regno Unito, in Austria, anche in Romania, lei oggi non sarebbe più seduta su quella poltrona; sarebbe stata mandata a casa, perché troppe sono state le circostanze che l'hanno vista incapace di svolgere il suo ruolo. Le vorrei soltanto ricordare il disastro che ha fatto quando in occasione dell'assalto alla CGIL, CGIL, lei non riuscì a fermare un signore, Giuliano Castellino, che era un sorvegliato speciale con obbligo di residenza e divieto di partecipare alle manifestazioni. oltretutto che lo stesso signore - si fa per dire - da piazza del Popolo un'ora e diciassette minuti prima disse: andiamo tutti alla CGIL a prenderci quello che è nostro. Lei ha risposto ha risposto che non poteva fare niente, perché se l'avesse fermato sarebbe successo qualcosa di peggio. Il peggio però non poteva essere, perché lei, signor Ministro, ha raggiunto il peggio dell'operato del suo Ministero.

60.000 rispetto i 10.000 di due anni fa. Lei si fa qualche domanda o sa solo leggere ciò che i suoi uffici le presentano per venire in Parlamento a dire cose che rimarranno nella storia di questa Nazione, quando in quest'Aula, alla domanda precisa su cosa faceva quell'agente in borghese quando spingeva quel furgone, sempre nel corso dell'assalto alla CGIL, lei rispose stava verificando la forza ondulatoria esercitata sul mezzo? Per quanto tempo dovremo ancora sentire queste risposte in un'Aula delle istituzioni? Lei pensa veramente che noi siamo ciechi e sordi? Lei pensa veramente che se dei Ministri in altri Paesi avessero avuto il tuo comportamento oggi sarebbero ancora seduti su quella poltrona?

Dico subito, prima di entrare nel merito dell'audizione, che fa bene a rivendicare il fatto di aver garantito, in una fase tanto difficile come quella in cui siamo e come quella che abbiamo alle spalle, lo svolgimento pacifico della stragrande maggioranza delle manifestazioni, sapendo quanta tensione c'è stata e continua a esserci nel Paese.

quanto successo nelle manifestazioni di cordoglio e di protesta per la morte di Lorenzo. Credo sia giusto farlo.

Se invece serve all'ennesimo attacco gratuito contro la Ministra dell'interno, contro il Governo, totalmente gratuito, facendo finta di dimenticare quali sono le diverse responsabilità che ci sono sulla gestione delle piazze, francamente questa discussione rischia di non servire a nulla.

Credo che questi siano davvero i principi cui dobbiamo ispirare la nostra riflessione e la nostra azione politica. Condivido, lo dico subito, anche la preoccupazione per le frequenti presenze di gruppi organizzati che si infiltrano nelle manifestazioni, condizionandole. La nostra La nostra condanna è totale, la nostra solidarietà alle Forze dell'ordine è totale di fronte agli attacchi di queste persone. Questo non è in discussione. Chi usa la violenza, va fermato e allontanato dai cortei. Signora Ministra, detto questo però, come lei sa meglio di me,

Occorre garantire la possibilità, per chi vuole, di manifestare pacificamente. Questo è il compito dello Stato, delle Istituzioni e delle Forze dell'ordine, evitando di coinvolgere, come purtroppo accaduto, giovani inermi negli scontri. La presenza di gruppi di facinorosi, di gruppi organizzati, non può giustificare quanto successo e che ha coinvolto giovani inermi. Insisto: lo Stato deve garantire la possibilità di manifestare in sicurezza.

poche manifestazioni. Questo però non vuol dire che non dobbiamo porci il problema; non si sono create le condizioni per consentire una manifestazione serena e pacifica a chi voleva farla. Su questo serve ragionare e capire. Su questo, mi pare l'abbia accennato quando ha parlato della consegna alla magistratura dei filmati, vanno accertate le responsabilità. Nel caso vanno presi provvedimenti anche rispetto a errori di valutazione che chi aveva la responsabilità della piazza doveva prendere. La nostra preoccupazione è che non si considerino questi incidenti di percorso o danni collaterali. Sono fatti gravi che occorreva evitare, che andranno evitati e che, forse, potevano essere evitati. Signora Ministra, lei ha fatto un'informativa molto onesta. Quando diciamo che c'erano informative, precedenti alle manifestazioni, che segnalavano che quelle manifestazioni erano attenzionate dall'iniziativa di gruppi che volevano creare incidenti, forse dobbiamo chiederci perché non siamo stati in grado di prevenire. Abbiamo di fronte una situazione sociale, una situazione sociale, legata anche al Covid-19, molto seria, che può generare tensioni. Quindi, serve prevenire, disinnescare lo scontro. Questa è una responsabilità che abbiamo tutti: chi controlla, chi ha la responsabilità dell'ordine pubblico, chi, come noi, ha la responsabilità di non farsi sommergere dalla propaganda e con quella accendere gli animi o

Non può e non deve passare l'idea, soprattutto tra questi giovani, di uno Stato nemico, che punisce il dissenso. Non è così. Quindi, signor

stanno dalla stessa parte delle Forze dell'ordine. Le Forze dell'ordine e le Istituzioni stanno dalla stessa parte degli studenti, anche quando gli studenti protestano. Questo è il principio su cui dobbiamo lavorare. Sta a lei, a noi, ai vertici delle Forze dell'ordine mettere in campo gli strumenti più adatti perché, in futuro, si possano contrastare efficacemente i gruppi di facinorosi, i gruppi organizzati, i gruppi che cercano incidenti, al fine di garantire a chi manifesta pacificamente di farlo in sicurezza, così come è giusto farlo in un Paese democratico che funziona e in cui le istituzioni funzionano come nel nostro.

In particolare sulla questione che riguarda gli studenti, io vorrei ricordare qui, a me stessa per prima, che quelli erano ragazzi che stavano manifestando

in piazza per manifestare - la Costituzione ne è garante - in una situazione anche molto difficile

il nostro dovere qui, come legislatori, è fare in modo che a quel disagio si risponda con fatti veri: è questa la vera discussione e il nostro compito. Questo però fa capo anche al Governo.

non partire dal dolore e dallo sgomento per la morte di Lorenzo Parelli: alla sua famiglia, a tutti i ragazzi che con lui hanno condiviso un percorso di scuola e di istruzione e speravano in un futuro di lavoro va il nostro pensiero e la riflessione più generale, che non è estranea a questa discussione, sull'inaccettabile vicenda delle morti bianche e di quanto accade, che nei giorni scorsi anche il presidente Mattarella ha ricordato, in quell'elenco importante di argomenti e impegni morali, sociali e legislativi che ha collegato alla tutela della dignità della Nazione. Quindi, ci sono varie questioni in questa informativa e non si può non partire dallo sgomento per la vicenda che poi ha innescato le manifestazioni e tutte le iniziative conseguenti. Però le cose vanno tenute distinte, perché non è che una tragedia drammatica, innegabilmente gravissima, può giustificare poi una serie di atti e di comportamenti. che vi sia lo segno e la rabbia e dobbiamo anche capirlo: è un sentimento di ribellione e di protesta che fa parte della vita sociale e della comprensibile indignazione di tutti. Quindi, che gli studenti abbiano assunto delle iniziative è assolutamente comprensibile; comprensibile; anzi, se non ci fosse una reazione di fronte a fatti di questa natura, ci sarebbe da interrogarsi su una società cloroformizzata dai *social*, da un modo di vivere che a volte sembra condizionato quasi più dalla comunicazione che dalla vita reale.

il Ministero dell'interno; che è parte rilevante dello Stato e lei, Ministro, lo sa perché lo ha vissuto in tutti gli aspetti. Quindi, anche se c'è il caporalato e forme di sfruttamento del lavoro, non è solo il Ministero competente per materia ma anche il Viminale che deve agire e operare, con le prefetture e sul territorio. A volte si dimentica che il Ministero dell'interno è lo Stato nella sua più operativa e rischiosa delle funzioni. Fare il Ministro dell'interno è una cosa - lei lo ha imparato - rischiosa scomoda, perché ci sono molte responsabilità che ricadono sul Ministro dell'interno e altre che non ricadono fisicamente sul Ministro ma che politicamente lo coinvolgono. Non sto qui a fare l'elenco delle questioni delle quali abbiamo discusso, dai *rave party* all'emergenza sbarchi: ci sono mille problemi che tutto il Governo dovrebbe affrontare insieme al Ministero dell'interno. Rimanendo sul sul tema della sua informativa, penso che sulle questioni del contrasto all'immigrazione clandestina e della sicurezza del Paese anche il Presidente del Consiglio dovrebbe dedicare più attenzione e più sostegno al Ministero dell'interno

Se abbiamo un Presidente del Consiglio così autorevole in Europa, metta a sedere tutti quelli che, appena c'è uno sbarco, girano la faccia dall'altra parte o si dimenticano che le navi sono spagnole, tedesche, sono dei Paesi che dovrebbero prendere le persone. le offriamo degli argomenti da far valere anche in Consiglio dei ministri. Sulla questione specifica, lei faccia tutte le verifiche del caso. Il Gruppo Forza Italia ha massima fiducia nelle Forze di polizia: nella Polizia di Stato, nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di finanza, nella Polizia penitenziaria. Ci possono essere stati errori? È possibile, in una gestione faticosa e difficile. Se ce ne sono, lei li verificherà e darà le istruzioni giuste. La proporzionalità dell'azione è un criterio fondamentale per chi gestisce l'ordine pubblico. Una manifestazione di ragazzi che escono dalla scuola è una cosa diversa da quella dei cosiddetti centri sociali che anche in questa vicenda hanno avuto occasione di fare violenza *(Applausi)* e di spaccare teste. Ministro, ha fatto un elenco, ma quanti sono stati i poliziotti e i carabinieri feriti in Val di Susa in questi anni solo perché si deve fare una ferrovia più moderna? Qual è il prezzo che stanno pagando poliziotti e carabinieri? C'è un bollettino. Ho sentito che lei citava Askatasuna (spero di averlo pronunciato bene). Quando sarà chiuso questo centro di violenza che in Piemonte sta aggredendo le Forze di polizia da anni e anni? Bisogna chiudere qua, bisogna chiudere là. Lo scioglimento: abbiamo detto di sciogliere tutto quello che va sciolto dopo i fatti che si sono verificati a Roma. Però anche queste cose qui perché devono avvenire? avvenire? Tutte le verifiche vanno fatte e noi pensiamo che a Roma e altrove anche le prefetture vadano valorizzate ancora di più, al di sopra delle questure o dei comandi territoriali delle Forze di polizia, affinché abbiano al loro vertice persone assolutamente adeguate e competenti. Però parliamo del personale delle Forze di polizia: diamo la solidarietà a chi è stato vittima di una tragedia enorme; comprendiamo che gli studenti possano avere rabbia, ma non i professionisti della violenza, tipo quelli dei centri sociali che si infiltrano nelle manifestazioni; non sono gli studenti indignati ma professionisti della violenza e dell'aggressione al popolo in divisa. *(Applausi)*. Questo va detto, colleghi, senza ammiccamenti ed equivoci. In questi giorni ho letto le note di tanti sindacati di Polizia: quelli del SIAP, del SAP, del COISP, del SIULP, di Italia Celere, che è un sindacato più piccolo fatto da quelli che stanno per strada a fare il lavoro in prima linea. Abbiamo collaborato con il Governo - il nostro Gruppo Forza Italia ne è orgoglioso - perché nella legge di bilancio si stanziassero risorse per le assunzioni e gli straordinari delle Forze di polizia. Ripeto, siamo orgogliosi di averlo fatto in questo Senato della Repubblica,

il tizio del centro sociale denuncia il poliziotto o il carabiniere, questi si deve pagare - il senatore Damiani che era in Commissione lo sa bene - le spese legali, le spese sanitarie. Abbiamo avviato delle iniziative, d'accordo con il Governo, perché chi rischia

successivo. Quindi, vogliamo garanzie per questo personale. Ben vengano le telecamere sulle divise, anche perché spesso vediamo nelle televisioni o sui *social* l'immagine che fa comodo: si vede il poliziotto che reagisce ma non si vede chi casomai lo bastona un attimo prima. *(Applausi).* Si fa il montaggio e lo smontaggio Ricordo che anni fa, signor Ministro, c'era un dirigente che faceva l'ordine pubblico a piazza Indipendenza, quando fu sgomberato uno stabile rimasto occupato per anni. disse una parolaccia mentre stavano intervenendo e fu subito biasimato sui *social*: un funzionario che dice una parolaccia? Eppure, non facevano vedere che sulla testa di quel funzionario e dei poliziotti erano state lanciate bombole di gas di 10-20 chili dalle finestre di quel palazzo occupato. E allora anche l'uso delle telecamere serve da parte dello Stato per impedire l'uso strumentale e parziale di alcune immagini che vengono utilizzate - basta cancellarne alcune - per far vedere il carabiniere o il poliziotto cattivo che invece si sta difendendo e sta garantendo la sicurezza e la libertà di tutti. Non vogliamo alcun eccesso; nessun eccesso ci deve essere, ma neanche alcuna resa dello Stato alle ragioni della legalità e dell'ordine. *(Applausi).* Si può e si deve manifestare, questo è un Paese libero dove ognuno deve poter esprimere la sua voce, ma secondo le regole, che poi, in questi anni di condizione sanitaria difficile, sono state inevitabilmente - ahimè più stringenti. Anche la politica, anche noi vorremmo fare riunioni nei teatri, nelle sale e nelle piazze, come abbiamo sempre fatto. E allora, vigili su quel che può non aver funzionato, si conceda a chi vuol protestare ovviamente di farlo, ma non si faccia una strumentalizzazione contro le Forze di polizia, a cui vanno dati gratitudine, riconoscenza, mezzi economici, assistenza materiale e morale. Grazie, quindi, agli studenti che vogliono esprimere le loro idee pacificamente, ma grazie al popolo in divisa che rischia e ogni giorno viene aggredito per la tutela della libertà di tutti i cittadini.

siamo in quest'Aula perché il Parlamento ha ritenuto urgente che lei venisse a riferire su un'ulteriore vicenda dalla quale emerge una netta critica al suo operato. Ministro, lei sa bene che noi della Lega non abbiamo mai fatto e non faremo sconti a nessuno quando si parla di sicurezza e ordine pubblico, quando viene in qualche modo messo in discussione il lavoro delle Forze dell'ordine. La prima analisi che dobbiamo fare per approcciarci al tema in modo costruttivo e scevro di strumentalizzazioni è che ciò che tutti noi abbiamo visto non sarebbe dovuto accadere. Signora Ministro, lei è chiamata a coordinare le prefetture, a organizzare la gestione dell'ordine pubblico con lungimiranza; è chiamata a valutare i rischi di situazioni che possono diventare esplosive e a comprendere fin da subito come la sicurezza dei manifestanti vada tutelata evitando che frange violente possano infiltrarsi e lavorare da dentro, per raggiungere obiettivi che nulla hanno a che vedere con le pacifiche rivendicazioni sociali giustamente portate in piazza. Non permettiamo che una cattiva gestione possa essere lo strumento per attaccare le donne e gli uomini delle Forze dell'ordine nel compimento del loro lavoro. È chiaro che nella gestione della manifestazione di Torino, che per giunta era stata autorizzata come presidio statico, le cose non hanno funzionato nel modo giusto: è stato permesso che frange violente dell'insurrezionalismo anarchico e facenti capo ai centri sociali si siano infiltrate tra gli studenti. È ovvio che tutto ciò è stato programmato ed organizzato nel tempo, da quanto emerge dalle immagini questi movimenti erano ben inseriti all'interno della manifestazione e avevano organizzato nei minimi dettagli le modalità di provocazione per arrivare allo scontro. La squadra mobile chiamata a gestire l'ordine pubblico della manifestazione ha capito fin da subito la pericolosità di ciò che stava accadendo e come avrebbe potuto degenerare se non si fosse intervenuti in tempo per contenere i manifestanti. Prevenire che certi fenomeni possano accadere richiede una guida attenta e un'attività di *intelligence* che va strutturata e strutturata bene. Dopo i noti fatti di Roma, culminati nell'aggressione violenta della sede della CGIL, ci saremmo aspettati un'attenta valutazione dei rischi della manifestazione di Torino, anche perché a Torino abbiamo dei professionisti dello scontro, antagonisti con esperienze plurime e pluriennali di attacco alle Forze dell'ordine maturate per lo più in Val Susa, ma non solo. Senatrice Fattori - che ora non vedo altro che agenti provocatori: Askatasuna non poteva mancare all'appuntamento di piazza Arbarello, mai perdere un'occasione per attaccare le Istituzioni fisicamente, era una situazione troppo ghiotta. Ovviamente, si è presentata arrivando equipaggiata di bastoni, mattoni e altri oggetti contundenti che hanno provveduto a lanciare al momento opportuno per scatenare la reazione della Polizia. La garanzia della sicurezza dei cittadini e la gestione dell'ordine pubblico si ottengono con il lavoro quotidiano, significa intuire, addestrare e formare gli uomini e le donne delle Forze dell'ordine, dotarli dei giusti mezzi, valutare quali siano i mezzi di difesa più idonei e soprattutto monitorare e reprimere gli ambienti dove la violenza contro lo Stato si annida. Da quando abbiamo assunto la responsabilità di Governo, come Lega abbiamo sentito il dovere di stare al fianco delle Forze dell'ordine, di garantire loro la massima dignità nello svolgimento dei propri compiti, abbiamo lavorato per potenziarne l'organico e per acquistare nuove dotazioni che ne facilitino i compiti, come ad esempio il *taser* e la *bodycam.* Non affrontiamo quanto accaduto con superficialità, ve lo chiedo per cortesia, cari colleghi. Sapete tutti quanto il nostro Paese è stato ferito profondamente dagli scontri ideologici, dalle guerre di parte, dal terrorismo rosso e nero. Quando si banalizza riferendosi all'accaduto, parlando di manifestazioni di studenti, ci si dimentica come le pagine buie della contrapposizione politica sfociata nel terrorismo e nella violenza sono state scritte proprio partendo dai movimenti studenteschi. Proprio oggi ricorre l'anniversario della morte di un giovane ragazzo, Paolo Di Nella: era il 9 febbraio del 1983, l'ultimo atto di quell'orribile stagione degli anni di piombo, quando un giovane studente fu ucciso a bastonate da frange violente armate dall'odio di parte. Facciamo attenzione a quando si svuota il contenuto di quanto accaduto a Torino, facciamo attenzione a criminalizzare le Forze dell'ordine. Basta poco per far sì che una scintilla si trasformi in un incendio. Noi della Lega siamo per l'assunzione delle responsabilità, sia chiaro. Se un poliziotto sbaglia, deve pagare come chiunque altro. Andranno approfonditi i fatti, andranno riviste le immagini, bisognerà capire nei minimi dettagli cosa è accaduto. Questo deve essere assolutamente fatto in tempi brevi. I giovani studenti e i loro genitori, che si sono ritrovati in modo inconsapevole in una situazione di alto rischio, devono avere delle risposte, devono poter sapere quali errori e soprattutto da chi sono stati commessi. Ministro, mi creda, siamo consapevoli del periodo storico che stiamo attraversando. Comprendiamo quanto sia difficile garantire il rispetto delle regole e come sia complicato arginare le manifestazioni violente che ardono sotto la cenere delle restrizioni e delle sospensioni delle libertà costituzionalmente garantite dovute alla gestione dell'evento straordinario e senza precedenti della pandemia. Ministro, mi creda quindi quando le dico che per queste ragioni la sicurezza e l'ordine pubblico devono essere una priorità per il Governo. Non possiamo permettere fatti come quello accaduto domenica sera in Barriera di Milano, sempre a Torino, dove decine di senegalesi, in festa per la vittoria della Coppa d'Africa, hanno aggredito un'auto di pattuglia, costringendola alla fuga. fuga. Uno dei principali problemi è costituito proprio dalla mancanza totale di timore e rispetto delle divise e dalla quasi totale certezza di impunità per chi dileggia, sputa o aggredisce i tutori dell'ordine. come Lega vigileremo sul suo operato e cercheremo di indirizzarla al meglio perché in questo momento non ci interessano le strumentalizzazioni. Non vogliamo capitalizzare dagli errori un facile consenso politico; noi siamo al Governo perché vogliamo contribuire al bene del nostro Paese anche a quello di chi, per 1.600 euro al mese, mette quotidianamente a repentaglio la propria vita per garantire la sicurezza di tutte le persone.

tragedia ha imposto, ancora una volta, l'urgenza di affrontare con serietà e decisione il tema della sicurezza sul lavoro, perché sul lavoro non si può morire così, a diciotto come a sessant'anni. Come ci ha ricordato il presidente Mattarella, le morti sul lavoro feriscono la società e la coscienza di ognuno di noi perché la sicurezza di ogni lavoratore riguarda il valore che attribuiamo alla vita. Questa tragedia ha sconvolto tutti noi e soprattutto i coetanei di Lorenzo: ragazzi per i quali una morte così atroce è stata un macigno pesantissimo, perché ognuno di loro avrà pensato: potevo esserci io, poteva capitare a me. Di certo questi ragazzi, così indignati e addolorati per la morte di un loro coetaneo, non possono essere definiti provocatori. Ministro, qualcosa va rivisto se alle provocazioni di adolescenti arrabbiati si è arrivati a rispondere caricandoli con i manganelli. Possiamo tirare in ballo tutte le norme possibili, ma ciò non toglie che quelli fossero solo dei ragazzi. Me lo lasci dire, Ministro: quelli sono i nostri ragazzi. E se, come lei stessa ha dichiarato, si è verificato un corto circuito, dobbiamo fare di tutto affinché non capiti mai più. Le parole di Gabriele, uno degli studenti presenti a quella manifestazione, sono esplicite: «siamo consapevoli delle restrizioni vigenti per la sicurezza sanitaria, ma ci sono tempi burocratici e tempi politici. Quello che è successo a Lorenzo ha significato tanto per noi e avevamo la necessità di farlo capire con ogni mezzo necessario».

in questo momento in cui escono già pesantemente segnati dalla pandemia che li ha privati del tempo più spensierato nei loro anni più belli, li ha allontanati dagli amici, dagli abbracci e dalla spensieratezza e scaraventati nella solitudine, nelle distanze e nella paura di contagiarsi e contagiare. Sono i ragazzi che hanno pagato il prezzo più alto di questa tragedia. La pandemia ha messo a dura prova la loro salute mentale se l'incidenza di depressione e ansia fra gli adolescenti è raddoppiata, se sono aumentati del 30 per cento i disturbi del comportamento alimentare un recente studio dell'università Cattolica di Milano ci ha rivelato che il 2 per cento degli adolescenti pensa quotidianamente a morte o autolesionismo. Questi ragazzi così provati sono e restano il futuro nostro e del nostro Paese e oggi ci chiedono aiuto. E se non siamo riusciti a proteggerli dai danni legati alla pandemia, abbiamo certamente il dovere di ascoltare questo grido di dolore che si esprime anche con la ribellione. Quei giovani in piazza ci chiedevano non solo di essere protetti, ma di imparare a guardare il futuro con i loro occhi. Secondo i dati del World Economic Forum, il 65 per cento dei bambini che oggi frequenta la scuola farà un lavoro che non esiste. E noi siamo pronti? In che modo li stiamo preparando al futuro? Quanto spazio diamo alla loro creatività, allo sviluppo dei loro talenti? E allora davvero aiutiamoli questi giovani, innanzitutto con l'ascolto e con il confronto e non con i manganelli. Poi aiutiamoli a scrivere con coraggio il futuro che gli appartiene. Papa Francesco, durante la Giornata mondiale della gioventù, diceva che il compito più arduo e affascinante che è stato consegnato loro è stare in piedi mentre tutto sembra andare a rotoli, essere sentinelle che sanno vedere la luce nelle visioni notturne. Il nostro compito, invece, è quello di essere bravi ad alimentarle quelle fiammelle, tenendo accesa la luce dei loro sogni e costruendo con loro, con coraggio e con visione, una storia all'altezza di quei sogni.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

Presidente, colleghi, vorrei mettere a fuoco insieme un aspetto dell'importante discorso che il presidente Mattarella ha fatto nel giorno del suo secondo giuramento, quello che si riferisce alla centralità del Parlamento. Avrei voluto farlo nell'ambito di una logica che riconoscesse valore a tutte le cose che noi facciamo nel nostro lavoro parlamentare e che molto spesso cadono in sacco vuoto. Mi riferisco, per esempio, alle interrogazioni parlamentari. Non è possibile che l'unico tempo che il Parlamento prevede per rispondere sia quello del *question time*, il giovedì dalle 15 alle 16. Con questi ritmi è evidente che nessuno di noi riesce ad avere risposte dai Ministri; non è possibile. Ora, può sembrare una piccola cosa, ma l'interrogazione nasce da un gesto di attenzione che il parlamentare fa nei confronti del territorio, nei confronti non solo dei suoi elettori, ma anche di quelle che possiamo chiamare le persone, che in fondo guardano al Parlamento e registrano anche in questo il senso dell'inadeguatezza del Parlamento. Io mi chiedo se, dopo l'intervento del presidente Mattarella, non si possa allargare formalmente il tempo dedicato alle risposte alle interrogazioni.

non si può credere che resti, da qui alla fine della legislatura, un'unica ora alla settimana per rispondere alle interrogazioni di 315 senatori.

Io credo che centralità del Parlamento significhi anche riprendere in mano l'organizzazione dei tempi e degli spazi. Ringrazio e lo faccio nel solco di quanto ha detto il presidente Mattarella, quindi penso di avere un autorevole copertura alle mie spalle.

ha indirizzato ai suoi colleghi, chiedendomi di leggerla in questa sede: lettera ai colleghi medici. Continuano a dire che le cure domiciliari non funzionano, io però ne ho curati quasi 600 e non ho avuto nessun decesso. Non sono caduto nella trappola del paracetamolo, perché l'esempio di Bergamo, con anziani lasciati cuocere per giorni nel loro letto a marzo 2020 con solo paracetamolo e i camion carichi di bare, mi sembra abbia chiarito che la terapia era fallimentare. Ovviamente riceviamo continui attacchi e a livello governativo e dei grandi virologi c'è la completa censura a queste cure. Ultimamente un collega mi ha offeso pesantemente di fronte ad un'altra collega che è rimasta inorridita. Sì, ci sono rimasto male, poi so quello che valgo e ho abbastanza autostima e non seguo la linea dell'odio, neppure se mi provocate pesantemente. Non fa parte di me e mai lo farà, proprio non ci riesco. Molti colleghi discriminano, in barba all'articolo 3 del nostro codice deontologico, le persone vaccinate da quelle non vaccinate, nonostante nel corso dell'ultima pandemia chi aveva ricevuto anche la tripla dose di vaccino si è ammalato lo stesso. Perché tutto questo? Perché questa violenza e odio dilagante, quando cercare di lenire e curare dovrebbe essere la soddisfazione principale per un medico, al di là delle scelte del paziente? È scritto nel nostro codice deontologico. Vi prego, colleghi che credete ancora nel nostro giuramento, mettete da parte idee malsane, siate e siamo di esempio verso un mondo che sta prendendo una brutta deriva. Ascoltiamo anche l'altro che non la pensa come noi, con quell'amore con cui guardiamo nostra madre. È da noi che deve partire un nuovo cambiamento, che porterà finalmente luce ad un mondo paralizzato dalla paura. Il dovere della cura fatta con coscienza e amore deve rimanere. Quanti effetti collaterali da puntura vedo? Tanti, eppure non mi tiro indietro e cerco di rimediare anche non dormendo di notte. La vita è sacra, unica. Pensate veramente di sentirvi meglio se trattate un ammalato a scarpate, se continuiamo a discriminare chi non ha fatto l'iniezione di Stato? È questa la medicina italiana, quella dei pazienti scambiati come mostri infettanti? Così in basso siamo giunti? Ho visto una donna gravida, fragile, sbattuta in mezzo alla strada senza assistenza medica. Ho visto persone piangere nel mio ambulatorio soltanto perché venivano accolte col cuore. Siete pure protetti finalmente dal vaccino, pertanto quali paure albergano dentro di voi? Che cosa è rimasto dei nostri studi universitari? Che cosa è rimasto della nostra umanità, dei poeti o degli scrittori che, come Manzoni, hanno descritto la peste? Che cosa è rimasto della libera scelta? Quali sono le priorità della vostra vita di medici? Cosa vi aspettate dal futuro? Che medicina avete? Avete dei progetti? Siete contenti e soddisfatti di voi stessi? Di notte cosa sognate? Al di là delle scelte fatte da ogni cittadino italiano, la cura e la guarigione sono innanzitutto una soddisfazione personale da tenere dentro, quel sogno che avevamo sui banchi di scuola all'università quando dicevi: chissà se da grande riuscirò, con le mie mani e il mio cervello, a salvare qualche vita? Ritorniamo lì, riprendiamoci quel desiderio che ci hanno rubato, facciamo rivivere quel giovane studente dentro la corazza dura che ci siamo imposti.

che il 24 gennaio 2022 la procura di Terni, dopo quella di Roma, ha definitivamente archiviato le infamanti accuse di razzismo e antisemitismo iniziate il 20 gennaio 2019 per un *tweet* stati trentasei mesi di gogna mediatica, con articoli di stampa denigratori verso una persona che aveva speso oltre trent'anni della propria esistenza a tutela dei più deboli e indifesi, battendosi contro ogni discriminazione di razza, lingua o religione. Oggi il giornalismo ha trasformato quella che dovrebbe essere la pietra angolare della democrazia, la libertà d'informazione, in un tribunale mediatico speciale e in troppi casi in gogna mediatica. Sui *media* vengono espressi giudizi intimidatori con vocabolario da linciaggio in pubblica piazza. Giudizi lesivi non solo della dignità di chi è oggetto dell'attacco, ma anche dannosi per la reputazione di giornalisti che invece di consumare la suola delle scarpe fondano gli articoli sul sentito dire, il pettegolezzo, ricorrendo ad espedienti per colpire le vittime del linciaggio, arrivando a formulare calunniose insinuazioni senza alcun riscontro delle fonti, persino ipotizzando l'inesistente e diffamatorio voto di scambio sui candidati al Quirinale. La procura di Roma già il 5 febbraio 2020 aveva ritenuto che le parole da me utilizzate in quel *tweet* erano prive di espressioni offensive, non risolvendosi in alcun modo in attacco personale gratuito, inquadrandosi nel diritto di critica

collaboratore della RAI che con un articolo diffamatorio dal titolo «Il grillino Elio Lannutti è stato citato a giudizio per istigazione all'odio razziale» il 3 agosto 2021 sul proprio profilo reiterava la calunnia, arrivando a concludere il *post* in modo minaccioso: «ci vedremo in tribunale senatore». Nell'Italia che punisce onesti servitori dello Stato per premiare gaglioffi, faccendieri, lestofanti, manutengoli del potere, tra i primi posti per corruzione e tra gli ultimi per libertà di stampa, sull'accusa di odio razziale, costruita ad arte anche per impedire che professionalità ed esperienza maturata nel mondo bancario e finanziario potessero essere messe all'apice di una Commissione bicamerale, ci sono stati oltre 1.000 articoli e centinaia di *talk* in TV e solo tre articoli sui media per dare notizia dell'archiviazione delle procure.

il mio breve intervento vuole ribadire il significato profondo della Giornata mondiale per la lotta contro il cancro, svoltasi il 4 febbraio. Il cancro non è più il sinonimo di una condanna senza speranza o senza appello. Oggi per fortuna, pur nella realtà dura e difficile che la persona colpita da tumore vive quotidianamente, la diagnosi di cancro è l'inizio di un percorso irto di tante difficoltà, di sacrifici, di sofferenze fisiche e psicologiche, che però sempre più spesso permette di vedere una luce in fondo al *tunnel*: la guarigione. È importante ottenere un miglioramento della qualità della vita del paziente ed il suo reinserimento nelle attività sociali. Tutto ciò senza dimenticare il difficile *iter* e le mille problematiche che iniziano dopo la diagnosi e proseguono con il percorso terapeutico, fatto di farmaci con i loro effetti collaterali, interventi chirurgici, terapie fisiche e di tanti complessi esami strumentali. Il tema di questa giornata richiama l'attenzione sull'importanza della diagnosi precoce, degli *screening*, sulla necessità di eliminare le diseguaglianze e le disparità delle cure. *Closing the care gap*, eliminare la disparità delle cure. Questo è lo *slogan* scelto per quest'anno. Dare sempre più risalto alla corretta informazione, alle campagne di sensibilizzazione sull'importanza della prevenzione e poter raggiungere l'obiettivo di un accesso alle cure migliori, uguali per tutti. Occorre infine porre rimedio ai danni e ai ritardi causati dal Covid-19 che rischiano, ora più che mai, di vanificare gli ottimi risultati raggiunti dalla ricerca, dai progressi scientifici, dalle nuove tecnologie diagnostiche e dai progressi terapeutici. Quante sale operatorie sono state chiuse, quanti interventi chirurgici sono saltati o sono stati ritardati, quanti ambulatori sono stati soppressi. Tutto ciò, Presidente, purtroppo tralasciando il fattore tempo e la sua importanza. Occorre riprogrammare rapidamente, per poter rimediare almeno in parte al tempo perduto, un piano di recupero dell'oncologia per non avere, dopo la pandemia da Covid-19, una prossima epidemia di casi avanzati di tumore non più operabili o trattabili per i ritardi e le carenze nell'assistenza accumulatisi in questi due ultimi due anni. Signor Presidente, occorre unificare gli sforzi. Ognuno faccia la propria parte per ridurre l'impatto del cancro sulle nostre vite. *(Applausi)*.